Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 9 maggio 2008 Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 7 maggio 2008, ha accettato le dimissioni rassegnate il 24 gennaio 2008 dal Gabinetto presieduto dall'on. Prof. Romano PRODI ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.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

Inoltre, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 8 maggio 2008 adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato il dott. Gianni LETTA Sottosegretario dì Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.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

Comunico inoltre che, con lettera in data 12 maggio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri mi ha informato della nomina dei Sottosegretari di Stato, il cui elenco sarà riportato in allegato al Resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca: «Consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri». Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi. Signor Presidente, sono lieto di essere qui per consegnarle il testo delle dichiarazioni programmatiche del Governo che ho appena illustrato dinanzi alla Camera dei deputati.

Grazie a tutti. capire e approfondire. Spero proprio che dopo il voto degli italiani - che è stato secondo me chiarissimo - si sia trovata quell'alternanza che da tanti anni era auspicabile e si avvii veramente una legislatura in cui maggioranza e opposizione possano trovare un accordo, chiaro, trasparente, per quelle innovazioni che sono ormai condivise e che devono essere introdotte nella nostra architettura istituzionale per poter fare dell'Italia un Paese veramente moderno e funzionale. Grazie a tutti. Le consegno, dunque, signor Presidente, il testo delle dichiarazioni.*(Vivi

Ringrazio il Presidente del Consiglio dei ministri e prendo atto della consegna del testo delle sue dichiarazioni programmatiche, rese questa mattina alla Camera dei deputati.

La discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio inizierà al Senato nella seduta pomeridiana di mercoledì 14 maggio, dalle ore 16 alle ore 21,30, con prosieguo nella seduta antimeridiana di giovedì 15, dalle ore 9 alle ore 11,30. Per la discussione generale sono state ripartite tra i Gruppi otto ore. La replica del Presidente del Consiglio, prevista per le ore 11,30 di giovedì 15 maggio, e le successive dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno luogo con trasmissione diretta televisiva. Nelle due settimane successive l'Assemblea esaminerà i decreti-legge in scadenza: nelle sedute di mercoledì 21 e giovedì 22 maggio saranno discussi il decreto-legge sul pubblico servizio di trasporto aereo, nonché ove approvati e trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati - i decreti-legge in materia di tutela della segretezza del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie e in materia dì trasporti ferroviari regionali; nelle sedute comprese tra martedì 27 e giovedì 29 maggio, oltre ai provvedimenti eventualmente non conclusi nella settimana precedente, saranno esaminati i decreti-legge in tema di protezione civile e di attuazione obblighi comunitari, presentati alla Camera dei deputati. Per tutti i suddetti decreti si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Comunico che in data 7 maggio 2008 sono stati nominati i componenti della Giunta per il Regolamento, di cui all'articolo 18 del Regolamento del Senato. L'elenco sarà pubblicato nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso di proporre al Senato - ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento - la nomina di una Commissione speciale, composta di ventisette membri in rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, perché esamini i disegni di legge di conversione del decreto-legge presentato al Senato e dei decreti-legge presentati alla Camera dei deputati, non appena trasmessi. In conformità ai precedenti, la Commissione speciale, oltre ad avere competenza di merito, assorbirà le competenze di ogni altra Commissione in sede consultiva, anche in relazione agli eventuali pareri obbligatori, nonché della 1a Commissione permanente in materia di presupposti di costituzionalità e di requisiti di legge dei provvedimenti, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito. I Gruppi parlamentari, su richiesta della Presidenza, hanno già provveduto a designare i propri rappresentanti nella Commissione speciale, la composizione della quale sarà pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna. La Commissione speciale è convocata questa mattina alle ore 12, presso l'Aula della la Commissione permanente, per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari, nonché per 1'eventuale esame del disegno di legge n. 4, recante conversione del decreto-legge n. 80, in materia di trasporto aereo, ad essa assegnato.